recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria,

portano la responsabilità la maggior parte delle forze politiche presenti in quest'Aula: sicuramente le forze che sostenevano il Governo Conte che l'hanno approvato, ma, allo stesso identico modo, le forze dell'attuale maggioranza che l'hanno costantemente difeso. Anzi, possiamo dire che dalla destra, già quando si manifestavano i primi disastri di questo provvedimento, arrivavano richieste di difendere il superbonus*.* Meloni ha definito fondamentale il superbonus per la crescita, come Salvini, magnificandone gli effetti sulla crescita economica. In realtà, questo Paese, che parla sempre di destra e sinistra, dovrebbe riconoscere nel superbonus il provvedimento più di destra mai fatto nella storia repubblicana,

per dare soldi a tutti: in piccola porzione a chi ne ha bisogno e in enorme porzione a chi non ne ha bisogno e rifà la casa a spese di operai, infermieri e impiegati. Il sistema è sbagliato nel modo in cui è stato costruito e disastroso nel come è stato applicato, senza una previsione di spesa razionale, senza un limite e con modalità che, attraverso la cessione, hanno dato luogo alla costruzione di un mercato di fatto secondario dei crediti, dei crediti, con 15 miliardi di truffe. 15 miliardi sono ciò che serve per mettere a posto sanità e scuola per un anno e 160 miliardi ciò che serve per farlo per serve per farlo per dieci anni. Ma certo è molto più difficile mettere a posto processi complessi ed è ciò che non si riesce più a fare in questo Paese. E allora l'alternativa è sempre e solo dare *bonus* e mance: questa, sì, un'attività *bipartisan* in cui ci sentiamo tutti - anzi, in cui vi sentite tutti - estremamente versati.

Pensavate che fosse una scorciatoia per la crescita e certo ha determinato un po' di crescita, ci mancherebbe: se i *bonus* complessivi sono 220 miliardi di euro e vengono dati sotto forma di *helicopter money*, cioè a chiunque,

A molte di quelle anomalie, di quei disastri, si poteva mettere mano con i soldi del superbonus. Oggi la soluzione è una misura retroattiva, parziale, che non funzionerà. Ve lo dico perché abbiamo provato a farlo in altri casi, per esempio, con un provvedimento chiamato "spalma bollette", che voleva spalmare i contributi

saranno enormi e vedremo che quello che stiamo discutendo qui oggi si ridurrà sempre di più e bisognerà fare correttivi sempre di più. si lesionerà l'affidabilità dello Stato che, come al solito *ex post*, dopo aver fatto un disastro, mette mano e lo fa male. Tuttavia è chiaro (o forse non lo è, non lo so) che un credito,

Se da tutto questo dobbiamo trarre un insegnamento, è che ogni volta che si sceglie la strada della mancia, grande a piacere, alla fine i conti con gli effetti di quelle mance bisogna farli. Oggi parliamo di superbonus, domani parleremo dei tagli *una tantum* fatti dal Governo nella scorsa legge di bilancio, perché hanno rimesso in moto un meccanismo di clausole IVA (ve lo ricordate?) che vanno confermate, altrimenti si alzano. Questo provvedimento è figlio di quell'ansia di trovare risorse per confermare altri *bonus* sui *bonus* fatti prima e così sarà in una catena infinita di irresponsabilità, mancanza di serietà e - permettetelo - mancanza di competenza. Come far accadere le cose rimane il grande sconosciuto in questo Paese. Mi spiace ma questa soluzione tardiva è sbagliata, non funzionerà e noi non siamo pronti a sostenerla. Grazie, presidente ancora una volta siamo chiamati ad approvare una correzione del cosiddetto superbonus, un provvedimento assunto per la prima volta nel lontano 2020, quando eravamo nel corso della pandemia del Covid, che ha determinato pesantissimi effetti sulla vita delle persone e sulla salute pubblica, ma anche conseguenze economiche davvero disastrose. Nessuno nega la validità dell'idea di istituire un *bonus* che consentisse di riavviare l'attività edilizia, sostanzialmente ferma, anche allo scopo di migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni; nessuno nega che l'edilizia è in piena salute e riesca a trascinare tutta l'economia. Purtroppo, non tutte le buone idee riescono sempre ad essere trasformate in una legge altrettanto buona. Non aver individuato nel provvedimento del 2020 limiti precisi all'erogazione dei *bonus,* che sono stati quindi messi a disposizione di ogni proprietario di casa che avesse voluto beneficiarne, ha determinato effetti perversi per il bilancio dello Stato; forse sarebbe stato sufficiente individuare un tetto reddituale per i proprietari di casa, per evitare che la misura si trasformasse in qualcosa di incontrollabile. Ugualmente, non si può dire della circostanza che il *bonus*, il cosiddetto 110 per cento, sia stato una concessione eccessivamente generosa: non si era mai vista nella storia dei *bonus* una percentuale di contributo così elevata per interventi edilizi. È stato davvero incredibile, peraltro, che lo Stato non abbia potuto o saputo preventivare un costo finale del provvedimento, neppure per approssimazione, e sia andato avanti così alla cieca senza sapere quale fosse la meta finale. Inoltre, quando la misura del superbonus fu varata, non sono stati pensati controlli adeguati sulla presentazione delle richieste e, soprattutto e certamente, sui lavori. Da qui gli abusi sull'uso del superbonus, che hanno imposto ai vari Governi che si sono succeduti negli ultimi quattro anni di dovere approvare numerosi interventi riparativi. Quello di cui discutiamo oggi è l'ennesimo provvedimento riparativo che si spera sia l'ultimo e che riesca a porre uno stop all'enorme buco nelle casse dello Stato. Aver deciso, con questo decreto-legge, che i lavori eseguiti con il superbonus daranno diritto a una detrazione in dieci anni anziché in quattro anni è una misura per rimediare ai danni e per dare respiro al debito pubblico. Lo stesso vale per la stretta

Allo stesso tempo, auspichiamo che il Governo intervenga anche con campagne di stimolo sull'educazione alimentare. Non sarà certo solo con l'introduzione di una semplice nuova tassa che si impedirà l'eccessivo consumo di bevande zuccherate, specie da parte dei giovani. Bene, infine, lo slittamento di due anni della *plastic tax*; ci sarà tutto il tempo per approfondire anche questa idea, evitando di provocare danni all'economia. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole al decreto in esame da parte del Gruppo UDC-Coraggio Italia-MAIE. Signor Presidente, quello che stiamo esaminando è l'ennesimo intervento tampone per fare ordine nel disordine dei *bonus* edilizi. Ora, a me non interessa ripercorrere il modo in cui siamo arrivati a questo punto, anche perché tutte le forze politiche hanno avuto un comportamento ondivago. Basta ricordare che chi oggi denuncia il buco di bilancio, nella passata legislatura chiedeva addirittura che il *bonus* 110 diventasse strutturale. Questi continui cambi delle norme, questo aggiungere e sottrarre burocrazia hanno assunto una dimensione patologica. I cittadini non hanno più la convinzione di siglare un patto con lo Stato, ma di fare una scommessa sul fatto che nel frattempo lo Stato non cambi le regole del gioco. E ancora peggio va alle aziende, che in questi anni hanno dovuto correre a dismisura perché non sapevano quanto e come i *bonus* sarebbero durati e quindi hanno preso lavori anche quando erano certe che non sarebbero state in grado di rispettare i tempi di consegna. Hanno fatto assunzioni senza sapere se in futuro sarebbero state in grado di mantenere quei livelli occupazionali e, per bilanciare questa incertezza, hanno aumentato i prezzi, concorrendo alla crescita dell'inflazione. Oggi migliaia di imprese nel settore edile sono sul punto di fallire per via della situazione a dir poco paradossale nella quale sono precipitati: migliaia di euro di crediti fiscali in pancia e carenza di liquidità e bisognerà capire come queste costanti strozzature hanno inciso anche sulla qualità dei lavori e delle materie prime che sono state adoperate, non sempre le migliori, ma quelle più rapidamente reperibili sul mercato e quindi non in grado di garantire la massima resa dal punto di vista dell'efficientamento energetico. Per spezzare questo circuito vizioso serve allora tirare una linea, introducendo regole che contemperino le ragioni di spesa pubblica con quelle per ridurre i livelli di inquinamento del patrimonio immobiliare italiano. Serve, anche per andare incontro agli impegni europei, un piano in cui i *bonus* non sono oggetto di contrattazione in ogni legge di bilancio, ma vengono stabilizzati per un periodo non inferiore a dieci anni. Solo attraverso la certezza delle misure il mercato dell'edilizia potrà uscire dalla schizofrenia di questi anni, i cittadini potranno programmare con calma i lavori sulla scorta delle proprie disponibilità finanziarie e degli altri impegni economici che, come famiglia, prevedono di avere. Le imprese avranno gli elementi per decidere se espandersi e se fare nuove assunzioni. Il mercato delle materie prime avrà tutto il tempo per organizzarsi, eliminando le ricadute inflattive. Insomma, sia la domanda che l'offerta assumeranno una dimensione sana e non quella di un'enorme bolla sempre sul punto di esplodere con pesanti effetti anche sul mercato delle nuove case, su quello dell'erogazione del credito, sugli obiettivi di contenimento della spesa energetica. Ovviamente facendo tesoro dell'esperienza di questi anni, il *bonus* dovrebbe avere un importo massimo di spesa detraibile, in percentuale, che di certo non può andare a totale copertura delle spese sostenute, ma dovrebbe anche prevedere la riproposizione della cessione del credito, almeno per una volta, per consentire l'accesso anche a chi non possiede la capienza fiscale. Capiamo le difficoltà di gestione del superbonus, ma perché il Governo non ha ancora avviato una riflessione sulla riforma complessiva del sistema? Non dobbiamo dimenticare che, grazie agli strumenti di agevolazione delle ristrutturazioni edilizie, negli ultimi venticinque anni, il settore è molto migliorato. Un settore che - bisogna ricordarlo - scontava gravi problemi di lavoro in nero, di elusione e di evasione fiscale e che invece oggi è tra i primi contribuenti fiscali, oltre ad essere un settore centrale in termini occupazionali. Questo settore oggi va quindi sostenuto e tutelato. Come vanno tutelati gli obiettivi più generali legati all'ambiente, legati all'ambiente, ma anche al valore complessivo del patrimonio immobiliare che - non dobbiamo mai dimenticarlo - rappresenta il principale bene rifugio di milioni di italiani. Permettetemi infine una considerazione per chi ci ha pesantemente insultati. Noi siamo e rimaniamo una forza di opposizione, ma lavoriamo nell'esclusivo interesse dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, guardando non solo alle convenienze elettorali di oggi, ma anche al domani. Per fortuna, a differenza di altri, non siamo costretti a vivere nella *trance* agonistica della campagna elettorale permanente. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato nel corso del dibattito in Commissione e in Assemblea pregevoli riflessioni di natura tecnica, contabile e finanziaria.

siamo stati accusati di essere a favore di questo Governo. E allora quale intervento migliore della fiducia per dire forte e chiaro che noi siamo contro questo Governo. Noi non votiamo la fiducia a questo Governo e, anzi, rimarchiamo le divisioni interne di una maggioranza che in campagna elettorale permanente dimentica la propria componente liberale e si atteggia a populista; ogni riferimento a Forza Italia è puramente voluto. quindi a dire perché votiamo no alla fiducia e poi approfondisco le questioni legate alla *sugar tax* e al superbonus. Siete un Governo degli annunci, signor Sottosegretario; Siete il Governo che ha scambiato la «*Gazzetta Ufficiale*» con Twitter, abbiamo tre riforme della giustizia al mese. Tutte bellissime, per carità; Non c'è un atto su cui poterci confrontare sulla giustizia. Siete il Governo che dice di volere l'elezione diretta, prima del Presidente della Repubblica, poi del Presidente del Consiglio, e poi portate in Aula un testo che è illeggibile ed invotabile persino dai vostri. Ve lo sta spiegando il senatore Pera.

ci sta dicendo che, come aumentano gli stipendi in Italia, non aumentano da nessun'altra parte. È anche sfortunata la nostra Presidente, perché le arriva il *report* successivo e immediatamente le si fa notare come, a differenza di tutti gli altri Paesi, il potere d'acquisto reale in Italia è peggiorato. E se non credete ai grandi professori internazionali, fate un giro nei mercati rionali, non nei mercati finanziari. Insomma, siete il Governo degli annunci. Proprio sulle tasse avevate promesso una rivoluzione liberale, che io ho sempre guardato con favore. Dopodiché, vi segnalo che avete reintrodotto alcune accise che Draghi aveva tolto. Avete alzato l'IVA sui prodotti per l'infanzia, a cominciare dai pannolini; avete reso più difficile il ritorno dei cervelli dall'estero, aumentando le tasse. Persino sulla casa avete aumentato alcune imposte. Siete il Governo delle tasse: voi. *(Applausi)*. Come facciamo a votarvi? Non soltanto per una coerenza elettorale, ma perché siamo profondamente delusi dal vostro comportamento. Abbiamo chiarito è un dibattito politico in cui la verità non conta, perché basta votare un emendamento per diventare "la stampella". Del resto, questo è un Paese in cui le *leader* dei principali partiti si candidano per il Parlamento europeo dicendo che non andranno al Parlamento europeo. Si candidano per avere una prima serata a "Porta a dimostrazione che la politica europea non conta niente, perché vi candidate per andare in un posto dove dite da subito di non voler andare. Non farò nomi, solo cognomi,: Meloni, Tajani, Schlein, Calenda. questa follia della politica ridotta ad "*annuncite*" la vediamo anche sui provvedimenti: e vengo al decreto-legge superbonus. Primo punto: c'è la *sugar tax*. Non è una novità: nel 2020, il Governo Conte-*bis* introduce la *sugar tax*. Noi facciamo una battaglia, allora eravamo in maggioranza, chiedendo di rinviarla, perché siamo contrari ad un atteggiamento in cui, quando c'è un buco di bilancio, si aumentano le tasse. Nel caso specifico, è una misura odiosa, intanto perché la *sugar tax* colpisce imprenditori e consumatori, a cominciare dal Mezzogiorno d'Italia, che rischiano di perdere posti di lavoro. C'è, però, un atteggiamento per cui, alla deriva scarsamente liberale, si aggiunge la deriva da Stato etico. Si dice che lo zucchero fa male e quindi si aumenta la tassa sullo zucchero. Lo Stato qui decide cosa fa bene e cosa fa male e gioca con la pressione fiscale, non per cercare di rendere più competitivo il Paese, ma per colpire quei settori che lo Stato etico decide che devono andare fuori mercato. con un capolavoro politico, visto che lo zucchero è, da sempre, uno dei settori in cui l'Italia ha avuto una storia. Noi, su questa battaglia della *sugar tax*, ci siamo imposti contro il Governo Conte e contro il Governo Draghi. Quando abbiamo visto che il Governo Meloni stava facendo una cosa giusta, cioè stava rinviando l'entrata in vigore al 1° luglio, abbiamo annunciato che avremmo votato a favore, con la maggioranza. Poi è successo che è successo che un partito della maggioranza, Forza Italia, per cercare di ottenere il consenso sul superbonus, ha scelto di annullare la propria storia liberale e la propria storia *no tax*, decidendo di mettere in difficoltà la maggioranza. Noi, in questo caso, non siamo stati per il Governo: siamo stati, come saremo sempre, per le imprese e per gli italiani. Ci viene detto: ma voi siete la stampella. No, noi siamo quelli che, se c'è da dare una stampella, la danno agli imprenditori italiani, che pure non ne hanno bisogno, non ad una maggioranza nella quale il regolamento dei conti passa anche attraverso uno scandaloso e

non ha mai lesinato critiche al presidente Conte? Penso di essere nella *top ten*, forse nella *top five*. Non ho alcun dubbio, dunque, nel dire che ci sono molte critiche da fare, ma questo provvedimento, per me sbagliato concettualmente, come dicemmo allora, è un provvedimento che poi è stato mantenuto nei due anni del Governo Draghi ed è mantenuto da due anni dal Governo Meloni.

dopo tre anni e mezzo, non si sia intervenuti ci porta a porci qualche domanda o no? Il punto è che questa è una misura sbagliata a cui il Governo ha scelto di dare una risposta che, secondo noi, non è all'altezza della critica che il Governo ha fatto. Se infatti dite che questa è la voragine dei conti pubblici, luogo dovreste spiegare quanti Ministri hanno utilizzato il superbonus. Anche su questo punto è necessario fare chiarezza: quando Conte ha dato i ristori a tutti, io da conferenziere avevo diritto a un ristoro di 25.000 euro, ovviamente ho detto: "non lo prendo". Vi sembra immaginabile che uno come me prenda il ristoro? Diamolo ai pizzaioli, ai commercianti, alle persone che stanno male; è un fatto di serietà. C'era una legge fatta da Conte che io non condividevo e non ho preso il ristoro che mi spettava. Come mai tanti Ministri che ci vengono a raccontare che il superbonus è il male assoluto lo hanno utilizzato *(Applausi)* e poi non hanno la forza di dire con franchezza che questa norma va cambiata? Fatelo, se siete capaci, ma dopo due anni che siete al Governo, anziché continuare a lamentarvi di Conte, provate a dire qualcosa anche voi su quello che immaginate di fare. Ho finito, signora Presidente. La destra è abituata a confrontarsi con una opposizione che le dice: "Autoritari! Fascisti! Illiberali!". Questo tipo di accuse piace da morire alla destra perché può giocare la carta dello scontro ideologico. Quando trova un'opposizione non ideologica che afferma i principi dello Stato di diritto, ma contemporaneamente vi contesta sugli stipendi, sui salari, sulle tasse, voi andate in difficoltà, perché siete pronti a confrontarvi con i no-TAV, siete pronti a confrontarvi con i no-TAP, ma quando vi arrivano i no-tax che vi dimostrano che noi sulle tasse abbiamo realmente ridotto la pressione fiscale

Per questo vi diciamo che siamo alla vostra opposizione e ci stiamo proprio bene, ma allo stesso modo non accettiamo lezioni da quella sinistra che sulle tasse vagheggia la patrimoniale e non si rende conto che in questo Paese la pressione fiscale è fin troppo elevata. Quando c'è stata la possibilità

con il Governo. Anche perché gli accordi con la maggioranza, come vediamo sulla RAI, li fanno quelli che di giorno in Parlamento urlano contro la Meloni, e poi la sera, tra una trasmissione de «Il Fatto Quotidiano» e un "accordicchio" di potere, sono sempre i primi a mettersi d'accordo con questa maggioranza.

mostruoso a proposito di modifiche normative sugli articoli 119 e 121 della legge n. 34 del 2020, da quando è entrata in vigore. modifiche in quattro anni sono un numero che davvero crea caos non nella legge, ma nel rapporto con i cittadini, con le imprese, con chi tutti i giorni deve fare i conti per tirare a campare. In più si introduce

dal punto di vista dei controlli, ad esempio sulla questione delle facciate. Tutti hanno parlato di questo problema.

siamo di fronte al fatto che dobbiamo fare una discussione tra di noi. Dobbiamo intervenire o no sul patrimonio immobiliare di questo Paese?

sono tutte cose da fare. Sul recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico, se si dice che bisogna andare in questa direzione, bisogna stabilire quante risorse si mettono per intervenire su questo tema. È stato sbagliato il superbonus

siamo in campagna elettorale e bisognava fare una grande propaganda. Il problema è un altro: noi oggi - e lo dobbiamo dire - con questo provvedimento, che introduce la retroattività, daremo vita a molti contenziosi. Quindi, saremo chiamati un'altra volta a intervenire, perché le imprese e i cittadini interverranno su questo problema, perché questa cosa è

vicini alle elezioni europee, dovremmo tener presente che cosa dice l'Europa, che dà l'indicazione di intervenire sul patrimonio pubblico e privato, ad esempio sulla questione del contenimento energetico. Allora, sarebbe da fare una corretta valutazione

sappiamo tutti che il settore edile, nel momento in cui si interviene e si ristruttura, ha un effetto di trascinamento su altri settori, perché se metto a posto la casa normalmente

a una discussione su questo tema tutta ideologica, tutta caricata dal punto di vista ideologico e non analizzata nel merito, perché, se andiamo a vedere i dati di merito,

bisogna proprio dire questo: io penso che la *sugar tax* contribuirebbe a ridurre le spese sanitarie in futuro. Invece si pensa di spostarla in avanti, perché è una

in modo determinato che noi, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo convintamente contro. Nello stesso tempo, vi devo anche dire

ci costringa a ritornarci fra qualche settimana o fra qualche mese. Questa che viene fatta e che voi proponete è un'ulteriore toppa che non risolverà il problema e che, anziché chiudere il buco, aumenterà la voragine. ci troviamo nuovamente a parlare di superbonus, una misura partorita dalla creatività ideologica del MoVimento 5 Stelle, nata male e purtroppo finita peggio. Si tratta di agevolazioni fiscali che sono sfuggite al controllo della finanza pubblica e che preoccupano ovviamente il Ministero dell'economia, che deve mantenere il controllo sul bilancio dello Stato. Tale misura si basa su un pensiero folle: lo Stato dà ai cittadini il 10 per cento in più di quello che spendono. Un sistema mai visto sul pianeta. Questo fatto, unito alla crescita esponenziale dei prezzi, alle truffe e al meccanismo della cessione dei crediti, ha contribuito alla crescita abnorme del costo del 110 Doveva essere un aiuto alle imprese del settore dell'edilizia in crisi per la pandemia e doveva efficientare il patrimonio edilizio italiano. Invece è diventato un incubo per i conti dello Stato, per le imprese, per i professionisti e per i cittadini. Capiamo quindi le ragioni del ministro Giorgetti, che con questo decreto e le sue modifiche ha l'obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici. Dall'altra parte, però, dobbiamo rappresentare anche le ragioni di famiglie e imprese, dobbiamo coniugare l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese con quello di tenere ordine nei conti pubblici, per finanziare le importanti misure concordate nel programma di Governo. Una tra queste misure è l'impegno a non introdurre nuove tasse. Ed è proprio grazie all'intervento decisivo di Forza Italia che è stata rinviata l'entrata in vigore della *sugar tax* per un anno *(Applausi)*, una tassa sbagliata, nata, come il superbonus, al tempo del Governo Conte, che avrebbe ricadute negative sui consumi delle famiglie e sulle attività delle imprese italiane nel settore alimentare. Una tassa inefficace, perché l'aumento dei prezzi farebbe crollare i consumi, impattando negativamente sugli introiti IVA e facendo sì che lo Stato incassi paradossalmente di meno. Le proiezioni parlano di una riduzione delle vendite del 16 per cento, di 5.000 posti di lavoro a rischio, di un impatto negativo sul *made in Italy*, con una riduzione di acquisto di materie prime italiane stimata in 400 milioni l'anno. Infine, le tasse non educano. Diversi studi dimostrano che nei Paesi in cui è stata introdotta la *sugar tax* non ci sono risultati positivi sulla salute. Se vogliamo ridurre sovrappeso, obesità e diabete, dobbiamo investire su una corretta educazione alimentare, che cambi lo stile di vita errato. Insomma, una tassa inutile, che oggi abbiamo rinviato, ma che è da eliminare definitivamente. Ribadiamo fermamente il nostro "no" a nuove tasse. Torniamo però al superbonus, che non ha certo dato i risultati sperati. Sappiamo che gli immobili efficientati sono una percentuale risibile del patrimonio immobiliare italiano, meno del 4 per cento degli edifici residenziali, rendendo flebile l'effetto di efficientamento energetico degli edifici e minimo l'impatto sulla riduzione dell'inquinamento. Forza Italia è più volte intervenuta per aiutare le famiglie, le imprese, i professionisti, gli artigiani onesti e in buona fede, che hanno avuto la sola colpa di credere a una legge dello Stato e si sono trovati in mezzo al guado.

di quest'anno. Purtroppo l'aumento dei prezzi, erroneamente non previsto in fase di strutturazione della legge, insieme all'iniziale facilità con cui si otteneva la cessione del credito, hanno reso ridicola la previsione iniziale di 40 miliardi di euro, portando il totale degli investimenti ammessi, solo sul superbonus, a circa 123 miliardi creando quindi un serio problema ai conti pubblici. Ecco perché vengono introdotte nuove norme, più rigorose, per l'utilizzo dei crediti del superbonus e degli altri crediti fiscali, arrivando a introdurre un sistema che spalma i crediti in dieci anni. Proprio su queste detrazioni fiscali pluriennali, che sono state portate da quattro a dieci anni, abbiamo cercato di spiegare in Commissione finanze quali siano i problemi legati alla retroattività della norma. Le norme devono valere dal momento in cui sono approvate in avanti, non indietro. La retroattività crea danni e confligge con i principi fondamentali del diritto. La retroattività incrina la fiducia tra i cittadini e le istituzioni e riduce la propensione delle imprese a investire in Italia. Questa norma determinerà problemi che investiranno nuovamente famiglie e imprese, creando migliaia di contenziosi. Basta vedere le reazioni del sistema delle imprese, del sistema bancario, delle associazioni dei proprietari e dei professionisti del settore dell'edilizia. Prepariamoci doverosamente ad aiutare le imprese che verranno danneggiate e rischiano il fallimento e le famiglie che andranno in difficoltà. Meglio sarebbe stato rendere facoltativo Questo avrebbe permesso a tutti gli attori di regolarsi al meglio rispetto alle proprie esigenze. Questa differenza di visione sul tema della retroattività (sul quale avremmo preferito una maggiore collegialità nella maggioranza) non ci impedisce, per la profonda lealtà che caratterizza Forza Italia, di essere favorevoli al provvedimento nel suo complesso, sperando che questo sia l'ultimo decreto-legge che modifica le regole del superbonus. Adesso è ora di guardare avanti. Torniamo finalmente a un sistema di bonus che ha funzionato fin dal 1999, consentendoci di ristrutturare il patrimonio edilizio italiano, sostenendo l'economia del settore dell'edilizia in modo stabile e facendo emergere il lavoro nero, cui spesso, purtroppo, sono legati gli incidenti sul lavoro. Dovremmo sviluppare un sistema di bonus stabile nel tempo, che garantisca a imprese e cittadini una pianificazione degli interventi, soprattutto quelli di efficientamento energetico; pianificazione temporale che eviterà l'aumento dei prezzi, che invece ha caratterizzato il Dovremmo lavorare affinché l'efficientamento energetico sia percepito come un'opportunità piuttosto che come un obbligo, come vorrebbe parte dell'Europa. Dovremmo integrare con un grande piano di rigenerazione urbana gli investimenti privati con quelli pubblici, per rendere le città più a misura d'uomo ed ecosostenibili, un volano per la crescita economica. Su questo tema sta lavorando proprio in queste settimane l'8a Commissione. Chi si occupa di fantapolitica ha raccontato che la fiducia era stata richiesta per problemi di maggioranza. Sappiamo bene che è stata richiesta per i tempi stretti per arrivare all'approvazione definitiva. Sempre chi si occupa di fantapolitica attacca la candidatura del nostro segretario Tajani alle elezioni europee, che però da vice *premier* e da Ministro degli esteri sui tavoli europei ci sarà sempre,

per le mie poche proprietà del superbonus e pensate che non ho neanche le entrate da conferenziere. Quindi, stia tranquillo non si agiti. Ricordiamoci che Forza Italia ci mette la faccia, perché si presenta con il proprio simbolo, non come altre forze politiche, che criticano e poi non hanno il coraggio di presentarsi con il proprio. Certo che su alcuni aspetti di questo decreto abbiamo discusso molto e continueremo a discutere in maggioranza. D'altro canto, il Governo è appoggiato non da un partito unico, ma da più partiti con idee in molti casi simili,

fondato da Silvio Berlusconi sia la migliore alleanza possibile per governare il nostro Paese. Per queste ragioni, voteremo convintamente sì alla fiducia al nostro Governo.

Si interviene nuovamente per introdurre nuove restrizioni sui *bonus* edilizi, si limita la cedibilità dei crediti fiscali, si modificano le agevolazioni fiscali, si introduce per la prima volta nel sistema giuridico italiano una norma con effetto retroattivo e si riducono le detrazioni fiscali addirittura al 30 per cento, mettendo a questo punto le mani nelle tasche degli italiani, perché questo provvedimento

che era stata varata negli ultimi trent'anni; basata sul settore dell'edilizia, che ha fatto crescere, poi, in maniera indiretta, tutti gli altri settori, la si sostituisce con il nulla, con il deserto. Questa è la politica economica del Governo Meloni, un vero disastro che ha nomi e cognomi: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti.

delle previsioni di spesa) a oltre 100 miliardi di spesa. E voi ci venite a dire che noi abbiamo sfasciato i conti pubblici. Ma di che cosa state parlando?

che peraltro è stato recentemente rettificato dall'Istat per ben 50 miliardi. Si tratta di un errore di previsione madornale: avete sbagliato la previsione di 50 miliardi, una cifra *record*. Per

macroscopici: innanzitutto, il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, in cui, con l'annuncio della cancellazione imminente della cessione dei crediti d'imposta, avete alimentato la corsa all'accaparramento della misura, che molti molti Ministri e molti rappresentanti del centrodestra hanno utilizzato meglio e prima dei cittadini italiani. Avete anche sbagliato la contabilizzazione, perché i crediti d'imposta li avete qualificati come pagabili e questo è stato uno dei motivi dell'aumento del *deficit*. Tale errore è reso palese soprattutto dalla stessa cancellazione della cessione dei crediti d'imposta. Forse sarebbe stato meglio consentire la cedibilità controllata dei crediti d'imposta, che peraltro doveva anche avvenire con l'introduzione della piattaforma tecnologica che lo stesso Ministro ha annunciato. Mi chiedo però che fine abbia fatto questa piattaforma tecnologica, che è stata completamente dimenticata da tutti, soprattutto dal Governo. A questo punto, vi chiediamo perché non siete intervenuti prima per monitorare e quindi bloccare la cessione del credito: per incapacità o per negligenza? Lo vogliono sapere gli italiani. I risultati della vostra politica economica sono ormai chiari: l'azzeramento della crescita, il crollo della produzione industriale da oltre tredici mesi, il calo dei consumi e dei salari reali, che hanno perso il loro potere di acquisto del 4,5 per cento rispetto all'Europa; il crollo del potere di acquisto, la povertà assoluta, i tagli alle pensioni e alla sanità, l'incapacità a mettere a terra il PNRR e, soprattutto, l'aumento della pressione fiscale. Questo è ciò che avete fatto in questi diciannove mesi e parlate a noi di buco di bilancio. Ma dov'è il buco di bilancio, dato che nessuna istituzione, né nazionale, né internazionale, lo ha rilevato?

in questione di ben 17,6 punti rispetto al PIL e le entrate fiscali aumentate di 140 miliardi. Entrando nel merito di alcune tematiche del provvedimento in discussione, in particolar modo lo spalmacrediti, con questa misura dimostrate di avere mancanza di innovazione, perché andate a rispolverare una vecchia soluzione a voi cara, introdotta già dal Governo Berlusconi, quando, per fare qualche spicciolo di cassa nel 2008 e nel 2011 con riferimento all'ecobonus (all'epoca al 55 per cento), portaste la detrazione a cinque anni, per poi portarla a dieci anni. Ma non vi smentite. Se questi sono i chiari di luna, non vorremmo trovarci come nel 2012. Lo spalmacrediti costerà il 15 per cento dei crediti ancora in portafoglio e ancora nei bilanci delle imprese, questo è il taglio che voi fate.

caro, per il quale introducete una norma completamente diversa. Il tutto per allineare il DEF 2024 alla NADEF 2023, ma per recuperare 2,4 miliardi ci chiediamo se non sarebbe stato forse meglio, piuttosto che fare questa manovra correttiva, non tagliare

Adesso ci chiediamo come farete a recuperare 20 miliardi per confermare cuneo fiscale e riduzione fiscale. e riduzione fiscale. Innanzitutto, la cancellazione della remissione *in* *bonis* dimostra che la vostra pace fiscale e il vostro fisco amico sono stati veramente una pura presa in giro nei confronti dei cittadini e avete così disatteso anche questa promessa. il Governo ha deciso di porre la fiducia in maniera strumentale sul provvedimento, solo per nascondere la frattura all'interno della maggioranza e questo lo testimonia l'astensione di Forza Italia in Commissione con riferimento all'emendamento governativo sulla retroattività della norma. Concludo, signor Presidente. richiamando un detto popolare: siamo arrivati alla canna del gas, con questo provvedimento è questo che state dicendo a noi e al Paese e noi vi diciamo che senza soldi non si canta messa

non è stato facile, perché con il taglio del numero dei parlamentari le Commissioni hanno un margine molto ristretto. La Commissione finanze, che prende decisioni per miliardi di euro, ha un voto di margine. Si era margine. Si era proposto di aumentare il numero con un supplente, ma non abbiamo voluto, perché non si possono cambiare le regole in corso e non è corretto, quindi siamo andati avanti con le regole precedenti. Non è stato facile, poi, perché il Gruppo Forza Italia non solo si è astenuto sull'emendamento governativo, ma ha anche votato con l'opposizione alcuni emendamenti. Nonostante tutto e nonostante l'atteggiamento di Forza Italia, l'emendamento governativo è stato approvato e i lavori si sono chiusi in maniera ordinata, come relatore al senatore Giorgio Salvitti, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, come intendo ringraziare tutti i senatori e le senatrici che hanno partecipato ai lavori per l'alto senso delle istituzioni dimostrato, perché non era

questi margini così ristretti non vanno bene in Commissioni che decidono per miliardi di euro: un solo voto aumenta il potere di ricatto e il potere delle *lobby*. Veniamo al merito. Sulla chiusura della stagione folle dei superbonus edilizi arriveremo in conclusione.

La cosa non stupisce poi molto perché il PD è abbastanza abituato a mettere nuove tasse. Ricordo che l'ultimo Governo che ha aumentato l'IVA è stato il Governo Letta, l'IRAP è stata messa da Prodi e l'elenco sarebbe lungo, ma io non voglio annoiarvi. Comunque, nonostante tutto, con questo provvedimento vengono ancora sospese *sugar tax*, e *plastic tax*. Ciò non è stato per niente facile, non solo per le motivazioni che abbiamo esposto prima, ma anche nel nel merito. Ecco, per darvi l'idea, l'emendamento che ha sostituito gli emendamenti delle Forze di maggioranza, Lega e altre forze di Italia Viva, che proroga la *sugar tax*, vede tre righe di emendamento e due pagine di copertura,

e dà la misura della difficoltà che adesso ci troviamo ad affrontare. Altro che andare avanti a ballare sul Titanic. Noi, d'ora in poi, dobbiamo coprire con ulteriori entrate o con corrispondenti tagli di spesa. Veniamo però ancora al merito: c'è un'altra

È una norma importante. Finora i controlli ci sono stati e sono già emersi 16 miliardi. Figuriamoci, è una cifra enorme, ma è la punta dell'*iceberg*. I controlli attualmente sono solo documentali, quindi vengono fatti sui documenti, come può fare l'Agenzia delle entrate dal suo pc. È chiaro che è difficile andare in ogni casa,

Il cappotto c'è su quattro pareti, come dichiarato? Vediamo. Il cappotto è di 8 centimetri invece che 3? Basta fare un buco con il trapano. Si tratta quindi di cose semplici. cose semplici. La pompa di calore della marca x ha tale potenza? Basta leggere la targhetta. Ecco, è evidente che controlli di questo tipo possono essere fatti semplicemente da un vigile e da un geometra insieme e, a tappeto, porteranno giustamente a vedere quello che è stato fatto bene e quello che non è stato fatto bene. A tale riguardo sono state dette molte cose, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Servono competenze particolari? No, abbiamo spiegato che si tratta di controlli semplici, niente di trascendentale. che i proprietari non fanno entrare. Non lo so, se un proprietario non fa entrare, vuol dire che ha qualcosa da nascondere e quindi poi arriva gli l'Agenzia

dieci anni. Quindi, le cose basta volerle fare. Sulla fine della folle stagione dei *bonus*, era necessario dare uno stop definitivo: era necessario. Si poteva fare un altro giro di valzer sul Titanic, aspettando le elezioni, magari pensando di guadagnare qualche voto in più? Secondo noi, no. E ha fatto bene il ministro Giorgetti e ha fatto bene la Lega che, con alto senso dello Stato, hanno messo un punto, uno stop, e hanno detto basta subito. La serietà paga. Mi tocca citare un libro di Einaudi che ho sul comodino, perché questo passo si adatta perfettamente alla nuova stagione che dobbiamo abituarci tutti a vivere. Siamo al 16 ottobre 1920, ma sembra scritto ieri: "lo Stato seguita da anni a spendere più di quanto incassa. Finché durava la guerra e con essa la forza maggiore, il fatto era spiegabile". Finché c'era la pandemia, il fatto era spiegabile. Continua Einaudi: "adesso non c'è più. Ora non più. Bisogna cominciare a rimettere la casa in ordine dall'alto. Bisogna che lo Stato contragga le spese fino a farle rientrare nei limiti delle entrate. Noi non abbiamo il pareggio secco, però abbiamo un *deficit* da rispettare. Un privato che si ostinasse a spendere più dei redditi, sarebbe fatto interdire dai tribunali e messo sotto curatela". Einaudi Einaudi continua: noi non vogliamo che lo Stato italiano sia messo sotto la curatela di nessuno, nemmeno sotto quella della Società delle nazioni (oggi sarebbe la *troika*) e perciò vogliamo che esso non tardi a mettere in equilibrio il suo bilancio. Ecco, questo è quello che ha fatto il ministro Giorgetti; questo è quello che vuole la Lega. Qualcuno pensa che ballare sul Titanic paghi. Noi pensiamo che la serietà paghi.

quello di oggi è senz'altro quello politicamente più grave e più significativo e che probabilmente segna anche un cambiamento di fase per gli equilibri della maggioranza.

nelle mani, sulla testa e per il voto di singoli senatori. Io credo che queste affermazioni vadano sottolineate, perché sono gravi e importanti dal punto di vista del passaggio politico che stiamo vivendo e che sta vivendo la maggioranza. *(Applausi)*. In effetti, la giornata che abbiamo vissuto martedì scorso in Commissione finanze non può essere derubricata alla cronaca di una normale dialettica, di uno scambio di opinioni tra alleati e tra forze di maggioranza. È stato molto, molto di più. Signor Presidente, mi lasci però ringraziare il presidente Garavaglia, per l'equilibrio e la sobrietà con cui ha condotto una giornata che è stata lunga, faticosa, impegnativa ed anche rischiosa, per la maggioranza e soprattutto per il Paese. La maggioranza, infatti, ha traballato, e poi ha provato a salvarsi, con un *blitz* così politicamente sfacciato che il presidente La Russa ha dovuto bloccarlo, consapevole della portata politica di quel tentativo, al di là della legittimità procedurale. Infine, la maggioranza si è salvata, com'è noto, grazie, non alla farina del proprio sacco, ma a qualche aiuto da casa. La questione rilevante dal punto di vista politico credo però sia un'altra e vorrei usare questi pochi minuti per sottolinearla. La maggioranza è andata in difficoltà su una misura nata nel 2020 come intervento anticiclico, com'è stato ricordato da altri, che senza ombra di dubbio ha prodotto un impatto sulla crescita in una fase di grave recessione per il Paese dovuta al Covid-19. L'evoluzione di questa misura è stata gestita per quasi due anni da questo Governo e per un periodo un po' più breve da un Governo, quello guidato da Mario Draghi, sostenuto da due tra i tre partiti maggiori che formano questa maggioranza. *(Applausi)*. Questa maggioranza, con il ministro Giorgetti in testa, non è stata in grado di immaginare una *exit strategy* in tempi e modi tali da non arrecare danno a famiglie e imprese. Non è stata nemmeno in grado di rispondere ad alcune delle domande che noi, come Partito Democratico e come opposizione, abbiamo posto nel momento in cui è stato presentato e poi approvato il DEF. Ad esempio, perché il Governo Meloni-Giorgetti più di una volta ha prorogato in questi diciotto mesi le misure del superbonus, *in primis* una di quelle più contestate, ossia quella relativa alle abitazioni unifamiliari, le cosiddette villette? Non abbiamo ricevuto risposte a queste domande. Dei 122 miliardi contabilizzati nel DEF che valgono su quattro anni, quale sia la quota che va a cadere sulle annualità 2023 e 2024, per una più precisa contabilità dei costi e della costruzione del *deficit*, ma non è stato possibile avere risposta a questa domanda. Insieme a imprese e sindacati, abbiamo chiesto di sapere qual è la stima delle risorse che entreranno nel 2024 a valere sulle fatturazioni fatte negli anni precedenti, che quindi avranno un impatto sull'anno in corso. sono arrivate risposte convincenti dal Governo. Vorrei però sottolineare un altro punto. Ieri sono state pubblicate le previsioni economiche dell'Unione europea, che ci suggeriscono una riflessione anche di ordine politico che credo quest'Aula debba

per arrivare all'1,1 per cento nel 2025. Aggiungono gli analisti dell'Unione europea che questi pochi decimali di crescita sono dovuti prima agli effetti degli investimenti sostenuti negli anni passati nel settore dell'edilizia

Avevamo già detto in occasione della presentazione del DEF che i vostri numeri parlano chiaro: senza il PNRR, l'Italia sarebbe in stagnazione, se non in recessione. Che cosa vogliono dire politicamente queste considerazioni, ossia crescita sostenuta dai *bonus* edilizi e poi dal PNRR? Che il Paese in questi anni è cresciuto, anche quando è cresciuto poco, grazie a misure di politica economica che non sono farina del sacco di questo Governo *(Applausi)*, ma sono state pensate da altri Governi. Presidente, non abbiamo mai speso un minuto in quest'Aula a discutere di una proposta di politica economica che fosse frutto dell'elaborazione di questa maggioranza *(Applausi)*, dell'unità delle forze politiche che sostengono la *premier* Giorgia Meloni. Non è un caso che ci abbiate presentato qualche settimana fa un DEF politicamente muto, che nulla è in grado di dire su quale sia l'idea di politica economica di questo Governo. Sorge il dubbio che sia così muto perché le idee sono molto diverse e contrastanti. Qual è l'idea che sorregge questo Governo? L'autarchia agricola, che sembra emergere dalle parole del ministro Lollobrigida? La difesa delle rendite da posizioni acquisite, vedi la vicenda dei balneari *(Applausi)*, che sembra spingere le idee del ministro Salvini e di altri? Oppure la difesa degli interessi di famiglia che emerge dalle parole dei colleghi senatori di Forza Italia? O il ritorno all'*austerity*, sostenuto da Giorgetti, ministro dell'economia, che non è stato in grado di negoziare in Europa un nuovo Patto di stabilità più vantaggioso per il Paese? Forse il presidente Garavaglia, dalle ultime citazioni fatte, condivide questo approccio che guarda a una nuova *austerity*. Per queste ragioni, signor Presidente, al di là del merito, che noi abbiamo trovato sbagliato rispetto alla soluzione individuata in questo decreto-legge, con il grave *vulnus* della retroattività - è stato ricordato da altri colleghi - che non solo mette in difficoltà difficoltà imprese, famiglie e banche, ma lede un principio fondamentale di legittimo affidamento tra cittadini, imprese e istituzioni rispetto alla certezza del diritto - quindi siamo profondamente contrari nel merito - la soluzione - la soluzione si inquadra in un quadro di non chiarezza e di grande confusione sull'idea di politiche per la crescita e di politica economica che questo Governo porta avanti. Noi riteniamo che il nostro voto fermamente contrario anche al provvedimento di oggi sia uno stimolo indirizzato al Governo e alla maggioranza a far chiarezza, affinché giornate come quella che abbiamo vissuto martedì

che ha messo in questa fase *(Applausi)*, ma soprattutto per ultimo, ma non ultimo, il presidente Garavaglia per la spiazzante correttezza, per la lucidità e la flemma che ha tenuto in Commissione e soprattutto per la sua alta professionalità,

il nostro tempo e abbiamo lavorato tanto in Commissione. Abbiamo scelto di avviare un lungo e variegato ciclo di audizioni, audendo portatori di interesse, categorie, professionisti. Abbiamo accolto come maggioranza tutte le richieste di proposte di audizione pervenute dai Gruppi o dai singoli. Spiace, però, che ad aver assistito alle audizioni siano stati in pochi e sempre i soliti. Immagino però che i miei colleghi abbiano letto attentamente le memorie degli auditi. Ma spiace l'assenza in Commissione, perché avrebbero potuto ascoltare dal vivo la reazione degli auditi alla domanda del Presidente, che ha fatto in maniera puntuale a ogni singolo audito, fosse esso rappresentante di una categoria, un professionista o un portatore di interesse: bene, avete ragione; se ci aiutate a trovare la copertura, noi siamo disposti ad accogliere le vostre richieste. Quello che colpiva non era la domanda del Presidente, ma la reazione degli auditi: nessuna reazione, se non quella Voglio leggere a questo punto, affinché le mie parole siano certificate, parti della memoria della Banca d'Italia. Ci avete attaccato, a inizio legislatura, sul fatto che qualcuno di noi potesse non avere grandi rapporti confidenziali con la Banca d'Italia e, quindi, immagino che una memoria della Banca d'Italia su questo tema sia per voi quasi come la Bibbia per altri: «Sebbene le numerose modifiche normative appena descritte abbiano cercato» - cioè quelle avvenute dalla creazione ad oggi - «di limitarne l'entità, gli oneri e le finanze pubbliche sono risultati elevati e la loro stima è stata ripetutamente rivista al rialzo»; «A ciò si è aggiunta la mancata predisposizione di un efficace sistema di monitoraggio iniziale», non essendo sufficienti «quelli pubblicati mensilmente da ENEA, relativi allo stock dei soli lavori di riqualificazione energetica energetica asseverati. In entrambi i casi la normativa ha consentito tempi lunghi per le comunicazioni, rendendo arduo osservare tempestivamente le accelerazioni della spesa». Ovviamente salto alcune parti: «L'elemento dirimente per le decisioni è costituito dalla trasferibilità del beneficio». «Come già ricordato, tuttavia, la fruizione del Superbonus è stata consentita anche attraverso lo sconto in fattura da parte del fornitore e la cessione a terzi in alternativa alla consueta modalità diretta in dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario. Questa peculiare modalità di godimento supera di fatto il vincolo posto dalla capienza fiscale del contribuente e quindi aumenta la probabilità che l'intero beneficio sia utilizzato». classificazione statistica del Superbonus ha un impatto rilevante sul momento in cui la spesa si riflette sull'indebitamento netto, ma non sul debito pubblico, che in ogni caso ne risente man mano che si materializzano le uscite di cassa». Ho sottolineato altre parti e mi auguro che i colleghi abbiano la decenza

cento in più, rispetto al già tanto 100 per cento, mi sembrava tantissimo, oltre il troppo". Ma a voi oggi ancora, dopo la discussione generale e dopo le dichiarazioni di voto - è ovvio - sembra tutto normale e ben proporzionato, perché non vi rendete conto di quello che è accaduto in questi anni. anni. Avete perso tempo a magnificare "Giuseppi" - conosciuto così a livello internazionale - e a pensare alla grande opera per portare in Italia 220 miliardi del PNRR, di cui 150 (cioè i due terzi) sono una finanziaria, su cui paghiamo anche gli interessi. Oltre Oltre al PNRR, dobbiamo essere ricordati per qualche altra miliardata a carico dello Stato. Ecco il Gollum, il mostro: 219 miliardi di soldi dello Stato, della collettività, a pagare il vostro "gratuitamente". In questa magnificenza, intestatevi totalmente il 110 per cento e il superbonus. A noi il "gratuitamente", credetemi, non piace: "gratuitamente" - ve lo ricordo - perché è vero che Conte non era più al Governo, ma gratuitamente è la parola più usata da "Giuseppi" e a dirlo non ero io, non sono io, ma è "Omnibus", su LA7, il 20 settembre 2022, in piena campagna elettorale, lo spot più imponente mai visto a carico dello Stato. l'ardire di ricordare - siano aumentate esponenzialmente le richieste. Certo, era già chiaro che noi avremmo guardato in maniera seria ai conti dello Stato e quindi quello spot creato quello che ha creato; una misura voluta da voi al 1000 per cento, vostra. La si sarebbe dovuta fermare prima, vi do ragione. Questo decreto sarebbe potuto arrivare anche prima. Il Gollum inarrestabile, che voi avete creato e che ancora non ha una forma, anche la Ragioneria dello Stato avrebbe dovuto stimare meglio ciò che avrebbe procurato. Ma la mente - non oso dire che mente che l'ha partorito è vostra; prendetevene la responsabilità, perché noi ci prendiamo le nostre. Cosa si sarebbe potuto fare con 220 miliardi? Quattordici ponti sullo Stretto di Messina, strade, scuole, viadotti, dighe. Una mente lungimirante avrebbe realizzato il più importante piano infrastrutturale degli ultimi cinquant'anni, invece del "gratuitamente". *(Applausi)*. Il sistema Italia avrebbe cavalcato, per il bene della collettività, realizzando per essa ciò che mancava, a beneficio di tutti, dalle imprese ai privati, a ogni singolo cittadino, nel ruolo che ricopre nel nostro sistema Italia, contro il beneficio di pochi.

vi do anche l'inserzione su Booking, se ne avete bisogno - a 1.593 euro per cinque notti. È questa la differenza tra noi e voi: il bene di molti per pochi, per la collettività. Noi badiamo alla collettività. Comprendo che urlare "gratuitamente" sia stato più proficuo elettoralmente di un grande cantiere Italia. Siamo coscienti - come ho detto prima - che il Gollum è ancora senza forma. Siamo stati sentinella e ora ci mettiamo la faccia con questo decreto. Sicuramente è doloroso,

misura sia importante per le casse dello Stato. I conti pubblici, come hanno già ripetuto diversi colleghi, sono sempre più importanti del ritorno elettorale dei singoli partiti. Quindi senza paura, a testa alta, come Fratelli d'Italia, rivendichiamo questo decreto-legge nella sua interezza, negli emendamenti parlamentari, del Governo e del relatore.

stop dal 2025 a compensazioni e contributi per banche, intermediari finanziari e imprese assicuratrici; rate in dieci anni per 12 miliardi di euro di detrazioni; non cedibilità delle rate residue; attività di vigilanza dei Comuni;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

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

Presidente, signora Ministro, l'interrogazione di oggi riguarda, appunto, le erogazioni nei confronti dei soggetti affetti da grave disabilità. sa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024, con l'erogazione di risorse progressive proprio per il triennio. La legge n. 234 del 2021 ha anche stabilito il piano delle risorse da ripartire, sempre per il triennio, stabilendo altresì che le Regioni concorrano con proprie risorse all'erogazione di prestazioni monetarie e anche dei servizi di assistenza diretta.

in vigore a partire da giugno 2024. Questa riduzione è stata motivata con la volontà da parte della Regione di aumentare il livello delle prestazioni dei servizi di assistenza diretta. Tuttavia, a fronte della decisione della riduzione dei contributi monetari diretti, non c'è stato un pari incremento dei servizi di assistenza diretta. quindi una platea di circa 7.000 soggetti affetti da disabilità grave o gravissima che saranno probabilmente danneggiati da una riduzione del contributo monetario, al quale non farà fronte un'assistenza diretta di tipo migliorativo. Stiamo parlando di una platea estesa, di circa 7.000 persone. L'interpretazione fornita dalla Regione per attuare questo taglio fa riferimento all'articolo 164 della legge 234 del 2021, ma noi riteniamo che questa interpretazione sia errata, perché effettivamente l'articolo 234 consente questa riduzione nei confronti delle persone non autosufficienti *over* 65, non di quelle non autosufficienti affette da disabilità grave o gravissima. Le chiedo, signora Ministro, se non intenda intervenire con riferimento all'interpretazione di questa disposizione nei confronti delle Regioni e se non intenda intervenire anche al fine di scongiurare che le Regioni, a fronte dell'incremento delle risorse del fondo, provvedano poi alla riduzione contemporanea degli aiuti umanitari diretti, che si traduce in un'assistenza minore, perché ci sono meno risorse anche per poter fare ricorso a interventi specifici. PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti e rispondo con gli elementi che mi sono stati dati dal Ministero delle politiche sociali che, come sapete, è quello competente sia sul Fondo nazionale per le non autosufficienze, sia sul Piano nazionale per la non autosufficienza. Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 rappresenta il risultato di un lungo lavoro di confronto, che ha attivamente coinvolto nella stesura la rete della protezione e dell'inclusione, con la partecipazione quindi di tutte le istituzioni interessate a livello centrale e locale. Nello specifico, il Piano si pone l'ambizioso obiettivo di raggiungere, in modo graduale e progressivo, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio. Al riguardo, il Piano nazionale per la non autosufficienza, nel proseguire il percorso virtuoso delineato dal legislatore nella legge di bilancio del 30 dicembre 2021, all'articolo 1, commi 162 e 164, mira a realizzare gradualmente un sistema non più basato sui trasferimenti monetari, ma sull'erogazione e sulla costruzione di un solido sistema di servizi alla persona. Corre l'obbligo di precisare che tale scelta non vuole rappresentare una diminuzione di tutele e di garanzie alle famiglie, ma anzi vuole determinare la costruzione di un processo in grado di sostenere meglio e più efficacemente i nuclei familiari e i diretti beneficiari dei servizi. Con la pandemia da Covid-19 è stata infatti palese la fragilità dei servizi sanitari e sociali di fronte ad un'importante emergenza, rendendo manifesta la necessità di pervenire al riconoscimento di una nuova attenzione e ad un nuovo rilievo nella gestione dei servizi dedicati ai cittadini tutti. Il potenziamento dei servizi territoriali riveste un ruolo fondamentale nel sostenere le categorie più vulnerabili ed è con questa visione che si vuole impostare la transizione verso una maggiore sicurezza nella possibilità di fruirne anche da parte delle situazioni in difficoltà. Quanto sopra rappresentato costituisce la chiave di lettura relativa allo sforzo di attuazione della costruzione di un sistema di servizi che, proprio in considerazione delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, è volto a mantenere l'erogazione monetaria, favorendo progressivamente, al tempo stesso, l'implementazione dell'erogazione dei servizi con un carattere graduale che rispetti pienamente le platee di riferimento. Tale impostazione è stata mantenuta e ulteriormente rafforzata con l'approvazione in via definitiva del decreto legislativo n. 29 del 2024, attuativo delle previsioni della legge delega n. 33 del 2023 sulla non

chi ha partecipato alla stesura della carta dei diritti delle persone con disabilità dell'ONU e della successiva, un po' tardiva, ratifica in Italia, sa che un elemento fondamentale è quello dell'attenzione per le donne, per fortuna, perché rivendichiamo e rivendico una differenza sostanziale nei pregiudizi, nell'elaborazione dei servizi e nella prospettiva di scelta di vita e anche di scelte sulla sessualità, come poter generare o no vite. Certamente le barriere legate ai servizi di ginecologia e di ostetricia anche ai consultori familiari ostacolano questo percorso, già difficile in sé, anche perché abbastanza diverso da territorio a territorio nella nostra meravigliosa Nazione, lunga e stretta, ma con qualche differenziazione inaccettabile, che vorremmo superare. Credo, Ministro - ne abbiamo parlato con preoccupazione, ma anche con passione tante volte

Signor Presidente, ringrazio il senatore Guidi per portare all'attenzione un tema davvero importante. Intervengo sulla parte di mia stretta competenza, anche perché nell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità abbiamo operato proprio in questa direzione, portando all'attenzione il tema delle donne con disabilità non solo nel contrasto alla violenza di genere, ma per il rispetto della salute delle donne e soprattutto delle donne con disabilità, che, per poter raggiungere le strutture e i luoghi di cura, hanno bisogno di un'attenzione all'accessibilità universale, che, secondo i princìpi della Convenzione ONU, dev'essere garantita a tutti, a maggior ragione quando parliamo di luoghi che devono essere raggiunti per il benessere, la cura, la salute, ma anche e soprattutto per il contrasto alla violenza. Pensiamo quindi ai centri antiviolenza quei luoghi dove tante donne che danno la loro disponibilità nel volontariato prestano servizio anche per dare ascolto ai casi più difficili e complessi. Proprio per questa ragione, ragione, a novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo invitato all'Osservatorio nazionale sulla condizione di vita delle persone con disabilità il ministro Roccella, col quale è iniziato un proficuo lavoro di collaborazione anche tra i due osservatori. Noi al nostro interno abbiamo voluto creare un gruppo di lavoro specifico dedicato al contrasto alla violenza sulle donne con disabilità. Il gruppo si sta muovendo su tre linee di azione specifiche: la prima è focalizzata sui temi della sui temi della comunicazione e dell'informazione, perché anche questi sono temi molto importanti, legati proprio all'accessibilità; la seconda affronta il tema degli *standard* minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio; la terza è mirata alla predisposizione di linee guida sulla violenza di genere e alla formazione degli operatori. aspetti sono oggetto di questo confronto anche nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Per garantire l'accesso ai servizi, ivi compresi quelli sanitari, per le donne con disabilità e per contrastarne ogni limitazione,

alle attività e anche alle prestazioni private, che va affrontato in una prospettiva nuova per tutti. Quando si fa qualcosa, lo si deve fare per tutti. Il rispetto della salute vale per tutti, ma a maggior ragione dobbiamo occuparci di eliminare i limiti e le barriere, di qualsiasi natura essi siano, soprattutto nella cura della persona, della donna e della donna con disabilità.

faremo in modo di collaborare con gli Osservatori, con lei e il Governo e tra noi senatori per dare più salute e libertà alle persone con disabilità donne, ponendo l'attenzione anche sulla prevenzione: penso all'endometriosi, ai tumori al seno e a quant'altro.

versano in condizioni gravi. Per quanto riguarda i disabili gravi, circa un ulteriore terzo vive da solo e in condizioni di difficoltà e ha bisogno di sostegno e di aiuto per tutte le mansioni che la vita quotidiana gli impone. Il tema che oggi abbiamo voluto portare all'attenzione dell'Assemblea del Senato è quello, in particolare, di un tavolo tecnico che lei sappiamo ha istituito presso il Ministero, soprattutto sul tema dei *caregiver*, cioè i

La prima domanda che le formuliamo è volta a capire a che punto è questo lavoro, se state procedendo in maniera significativa e quali risultati sono stati

come partito di Forza Italia è quella di cercare di attenuare al massimo le divergenze sul territorio nazionale e in questo senso le chiediamo se questo tavolo sta lavorando anche all'elaborazione di una normativa nazionale che possa cercare di attenuare le differenze sul territorio, tra l'altro cercando di adottare, ove possibile, le buone pratiche che in alcune realtà sono state attuate e in altre magari sono Da questo punto di vista, le chiediamo in particolare se è stato attivato un nomenclatore tariffario nazionale, in modo da adeguare anche dal punto di vista economico le provvidenze che vengono erogate a fronte di questi operatori che sono particolarmente utili per persone in condizioni di disabilità grave.

delle questioni affidate e, quando termineranno i lavori anche del terzo gruppo, si procederà a un confronto sui temi emersi in seduta plenaria, in modo che l'esito dei lavori rispecchi appieno le esigenze e le aspettative della platea nel suo complesso. Ci sono dei nodi da sciogliere, ma spero che nei

Procedo ora con le risposte fornite dal Ministero della salute, che ci ricorda che i lavori per l'emanazione dei nuovi nomenclatori sono iniziati subito dopo l'entrata in vigore del DPCM LEA del 2017: sono stati particolarmente articolati, hanno subito numerose pause ed arresti e solo dopo un lungo *iter* istruttorio nell'agosto del 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe, dell'assistenza specialistica, ambulatoriale e protesica, come previsto dal citato articolo del DPCM di gennaio 2017. Tuttavia, per consentire un maggior lasso di tempo per l'adeguamento dei vari sistemi ai diversi operatori coinvolti nelle nuove tariffe, con successivo decreto interministeriale del 31 dicembre 2023 è stato stabilito che le disposizioni entrassero in vigore il 1° aprile del 2024. Da ultimo, l'entrata in vigore del provvedimento è stata posticipata al 1° gennaio del 2025 su richiesta delle Regioni.

Sappiamo che il Ministro è molto sensibile al tema, che ha un'esperienza professionale e tecnica in questo settore e, quindi, siamo convinti che seguirà i i lavori con il massimo impegno e la massima competenza. L'auspicio che, come Forza Italia, non possiamo che formulare è quello che al più presto si passi

Signora Presidente, signora Ministra, l'interrogazione presentata riguarda il decreto legislativo approvato lo scorso mese in attuazione della legge delega del 2021 in materia di disabilità. Emerge con evidenza un problema legato alle risorse necessarie a garantire una riforma, su cui abbiamo lavorato

sperare in un passo in avanti per garantire nuovi servizi alle persone con disabilità. Lei stessa ha fatto riferimento alla semplificazione del sistema di accertamento dell'invalidità civile e a nuovi strumenti di accompagnamento, come il progetto di vita, parlando di innovazioni che che rappresentano il cuore della riforma. Bene, Ministra, è proprio come dice e noi siamo stati i primi a batterci per questa riforma. Le famiglie con disabilità oggi in Italia sono più di 2,3 milioni e quindi si tratta di una legge davvero importante perché mira a razionalizzare, semplificare e rafforzare gli interventi a favore delle persone con disabilità. C'è un però che è la ragione per cui siamo qua a porre il quesito. Mancano nel decreto governativo le risorse per dare attuazione alla legge. Siamo davanti ad un film già visto pochi mesi fa, ad esempio, con il decreto per le persone anziane non autosufficienti; annunci roboanti, apertura dei TG nazionali che annunciavano 1.000 euro al mese per tutti gli anziani e pochi fatti, a volte bugie per nascondere la vostra insussistenza e la totale mancanza di risorse, tanto che assistiamo all'assurdità che le risorse necessarie per l'assunzione del personale dell'INPS sono prese dal fondo in favore delle persone con disabilità. Ciò è assurdo, perché le nuove assunzioni che serviranno a far funzionare le sperimentazioni

Anche sulle sperimentazioni emergono dal citato decreto alcune criticità rispetto al rinvio a successivi regolamenti sulla base di criteri indefiniti e forieri di diseguaglianze tra cittadini con le stesse esigenze e alla mancata previsione di qualsivoglia norma in materia di monitoraggio delle sperimentazioni. Quindi le chiedo, signora Ministra, se ritenga che le risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo siano sufficienti e chiedo anche di sapere se non ritenga necessario prevedere una qualche forma di monitoraggio delle sperimentazioni previste; attraverso quali strumenti lei intenda seguire le diverse fasi di attuazione della riforma e se esista uno scenario alternativo in caso di esito negativo delle stesse per evitare un dispendio inutile di risorse pubbliche.

epocale che, io continuo a dirlo, spesso non viene compreso, perché è una riforma molto complessa. Le risorse sono state messe a disposizione da chi negli anni scorsi ha approvato la legge delega, quindi dai precedenti Governi, e sono state messe sui diversi capitoli, incrementati da questo Governo. Sicuramente, con l'avvio della sperimentazione, sono più che sufficienti, anche con l'entrata in vigore a regime della riforma. Quello che davvero è importante capire, però, e che bisogna diffondere in tutto il territorio è la nuova visione, il nuovo sguardo, un approccio che dice come funziona il progetto di vita. Questo ancora non è abbastanza chiaro e su su questo dobbiamo lavorare, a tutti i livelli istituzionali e tutti insieme. L'approccio al progetto di vita non richiede più che la persona bussi a tutte le porte per avere delle risposte, ma richiede che immediatamente vengano attivati i servizi e le misure dell*'équipe* multidimensionale. Quindi, capite che è un cambio è un cambio di passo eccezionale, sul quale noi dobbiamo investire. Investiremo, già a partire da quest'anno, venti milioni sulla formazione, in primo luogo nelle nuove Province che dovranno essere oggetto della sperimentazione, che parte, dicevo, dal 1° gennaio 2025. Nel corso del 2025 si vedranno quali sono i nodi,

cambiano molti aspetti e molte cose. Sarà necessario seguire da vicino il processo e destineremo fino a due o tre esperti per ognuna delle Province che affronterà la sperimentazione, per seguire direttamente, caso per caso, tutto quello che succederà. Sono stati messi a disposizione altri 25 milioni di euro per

grazie a delle risorse aggiuntive, potremo garantire il servizio, in attesa che un domani ci possa essere davvero un fondo unico che superi le estreme frammentazioni, anche a livello globale, tra i campi sanitari, sociosanitari e sociali, per la messa a disposizione dei servizi e degli interventi in favore della persona. Quello che è importante dire è che nel progetto di vita la persona è centrale. È un progetto partecipato, perché parte dai desideri, dal diritto di scegliere di ogni persona, previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Questo può essere condiviso anche con la famiglia. È chiaro, ripeto, che si tratta di una riforma complessa. Già solo nel descriverla si può comprendere quanto è complessa, ma ci dobbiamo credere tutti, perché è l'unica occasione che abbiamo per scardinare tante prassi

serve una grande formazione per capire che tutto questo è possibile se ci crediamo e soprattutto è possibile perché ci ha creduto prima di noi, a livello istituzionale e politico, il mondo delle associazioni e delle famiglie. Glielo dobbiamo, nel rispetto della dignità e della vita di ogni persona.

certamente ci mettiamo tutto il nostro impegno. Ma è proprio per questo che siamo insoddisfatti della sua risposta perché, al di là di ogni spiegazione, rimane il giudizio negativo sulle mancate risorse per una piena attuazione della legge in favore delle persone con disabilità. Bisogna evitare giri di parole e guardare alla sostanza. Già il fondo per le disabilità è stato ridotto in legge di bilancio; adesso viene ulteriormente tagliato. Siamo preoccupati, perché parliamo di un tema sensibile, la disabilità, appunto, e di obiettivi che da troppi anni il nostro Paese attende. Le do un consiglio, signora anche se non me lo chiede: smettete di creare aspettative, che poi si rivelano un *bluff*, nelle persone più fragili della nostra società. Oggi promettete ai disabili un progetto di vita individuale, ma non ci mettete le risorse. Avete raccontato agli anziani non autosufficienti che avrebbero ricevuto tutti un bel contributo, ma arriverà solo per pochissimi di loro. Avete raccontato che avete registrato il record di finanziamento della sanità pubblica ed invece le liste d'attesa si allungano e chi non ha i soldi rinuncia a curarsi. Avete raccontato che la disoccupazione è in calo, ma quel che aumenta è solo il numero dei lavoratori poveri a cui non volete riconoscere un salario minimo. La scorsa settimana ci avete presentato un Documento di economia e finanza vuoto senza la parte programmatica e strategica, perché non avete idea di dove trovare le risorse per finanziare quel che è già previsto, figuriamoci il nuovo; quindi sarete costretti a tagliare ulteriormente servizi che temo siano proprio quelli rivolti alle alle persone più fragili. Signora Ministra, sa come la chiamo io la riforma senza risorse? Propaganda, e gli italiani si sono già stufati di sentirla.

(SVP-PATT, Cb))*. Signor Ministro, lo scorso 26 aprile il *leader* del Movimento identitario austriaco, Martin Sellner, ha annunciato per il successivo 5 maggio una cosiddetta colazione rivoluzionaria rivoluzionaria in Sud Tirolo con il consigliere provinciale Jürgen Wirth Anderlan. Anderlan è noto per le sue posizioni secessioniste nei confronti dell'Italia, per la sua xenofobia, per le sue campagne di incitamento alla violenza contro i politici che hanno gestito l'emergenza pandemica. Per le forti manifestazioni di protesta, Martin Sellner ha annullato l'incontro, annunciando tuttavia che presto terrà a Bolzano una conferenza pubblica per dare ancora più peso e visibilità alla sua presenza. Martin Sellner è il teorico della cosiddetta remigrazione, un piano di espulsione su larga scala dai Paesi di lingua tedesca perfino dei cittadini austriaci tedeschi di origine straniera. Il piano, che dovrebbe avere un periodo di attuazione decennale, sarebbe quello di individuare uno Stato modello in Nord Africa dove spostare fino a due milioni di persone. Martin Selner è una delle figure più pericolose dell'intera galassia neonazista e xenofoba, con una forte attività di proselitismo anche al di fuori dei confini austriaci. Come ha rivelato un'inchiesta giornalistica, lo scorso novembre ha tenuto in Germania un incontro a porte chiuse con esponenti di Alternative für Deutschland, in cui ha illustrato i vari passaggi del suo piano di pulizia etnica. Per queste sue attività, Martin Sellner è stato bandito dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dalla Germania e dalla Svizzera. Va poi ricordato che storicamente il Sud Tirolo è il campo di battaglia per idee neonaziste, provenienti dai territori di lingua tedesca, con suggestioni pangermaniche. Ricordo anche che, in una terra dove è stata faticosamente costruita la pacifica convivenza tra gruppi linguistici diversi, i temi identitari legati a questioni etniche sono vissuti con particolare sensibilità. Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, se non concordi sulla necessità di intervenire e quali misure intenda assumere sulla scorta di quanto già fatto da altri Paesi, per evitare che Martin Sellner possa venire in Italia per propagandare il suo folle disegno di pulizia e sostituzione etnica. PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, Signor Presidente, intanto voglio precisare che lo scorso 5 maggio non ha avuto luogo alcun evento in provincia di Bolzano a cui abbia preso parte l'esponente politico austriaco di estrema destra Martin Sellner. Il 7 maggio scorso si è svolto un *flash mob* dei gruppi consiliari SVP, PD, Civica, Verdi, Team K e Freiheitlichen, per dare un forte segnale di dissenso rispetto alle recenti esternazioni del consigliere Wirth Anderlan e alle sue dichiarazioni sulla insindacabilità delle proprie personali frequentazioni; presa di posizione critica peraltro già espressa sui *social* anche da sodalizi riconducibili all'antagonismo locale, che si sono spinti fino a chiedere l'estromissione dell'Anderlan dal consiglio provinciale perché considerato un pericolo per i valori democratici, dopo aver portato avanti una campagna elettorale xenofoba. Ciò posto, secondo quanto riferito dalla questura di Bolzano, non risulta preannunziata nel prossimo futuro nessuna visita del Sellner nella Provincia di Bolzano. La situazione, comunque, continuerà ad essere monitorata dalla questura e dal commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano per ogni eventuale necessità.

a Bolzano a fare un comizio molto più grande, dove potrà esprimere le sue opinioni davanti a un pubblico molto più vasto. vasto. Ora, come lei ha anche citato, noi ci siamo già confrontati con il fenomeno di Wirth Anderlan, che è andato in Austria a dire che tutti i politici sono banditi corrotti e che i politici che hanno fatto le misure anti-Covid non devono solo andare in galera, ma addirittura nelle miniere ai lavori forzati. a noi sudtirolesi democratici premerebbe evitare che vengano anche dall'estero persone che la pensano così e che disturbano le relazioni amichevoli amichevoli che nel frattempo abbiamo costruito tra i gruppi linguistici. Per quanto ne sappia, anche il presidente della nostra Provincia, Arno Kompatscher, le ha espresso la sua preoccupazione. Pertanto chiediamo che venga monitorata questa situazione e che, in caso, vengano prese misure simili a quelle già prese in altri Stati democratici, anche europei.

Grazie, Presidente. Signor Ministro, noi vogliamo richiamare la sua attenzione rispetto alla condizione degli italiani all'estero. Si avvicinano le elezioni europee e proprio ieri l'Istat ci ha ricordato come la partecipazione al voto, la partecipazione politica, sia in preoccupante calo, soprattutto fra i giovani. Mentre per gli iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nei Paesi UE c'è la possibilità di esercitare il diritto di voto recandosi presso ambasciate e consolati, nel caso degli iscritti all'AIRE di Paesi extra-UE questa possibilità non è riconosciuta. Dopo la Brexit, per esempio nel Regno Unito ci sono circa 500.000 italiani, come anche altri ce ne sono in Svizzera, che, per poter esercitare il diritto di voto, devono per forza ritornare nel nostro Paese. Con il costo salito ormai alle stelle dei voli aerei, questo significa conculcare, limitare e rendere più difficile il diritto di voto per questi cittadini. Noi pensiamo che sia possibile un provvedimento urgente che consenta agli iscritti all'AIRE dei Paesi extra-UE di esercitare il diritto di voto, esattamente come avviene per gli iscritti all'AIRE che risiedono all'interno dell'Unione europea, e questo siamo a chiedere a questo Governo.

utile approfondimento, anche tenendo conto di uno specifico ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024, che proietta però ogni valutazione in vista delle elezioni europee successive a quelle di quest'anno. Le questioni, anche sulla base di quanto riferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono molteplici. A legislazione vigente, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono partecipare dall'estero esclusivamente i cittadini italiani in possesso dell'elettorato attivo e residenti nei Paesi dell'Unione europea, che votano presso seggi appositamente allestiti dalle nostre ambasciate e consolati. I connazionali possono decidere, in alternativa, di partecipare alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti al Paese membro di residenza oppure di rientrare in Italia a votare presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, beneficiando delle agevolazioni di viaggio previste. Allo stato, la partecipazione al voto dall'estero, come lei stesso ha ricordato, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non è pertanto prevista per i connazionali residenti in Paesi che non siano membri dell'Unione europea, ai quali è comunque assicurata la possibilità di votare in Italia, beneficiando anch'essi delle agevolazioni di viaggio. La modifica auspicata dall'interrogante, riferita solo a Regno Unito e Svizzera, peraltro presenta profili di criticità prima di tutto su un piano di equità, in quanto si tradurrebbe in un trattamento differenziato e discriminatorio nei confronti dei connazionali residenti dell'Unione europea in Stati diversi da Regno Unito e Svizzera. D'altra parte, un'eventuale modifica della legge che permette a tutti i connazionali residenti all'estero (anche quelli in Paesi extraeuropei) di votare per le elezioni parlamentari europee andrebbe valutata attentamente anche nei suoi delicati profili organizzativi. Signora Presidente, signor Ministro, noi abbiamo citato come esempio il Regno Unito e la Svizzera, ma è evidente che questo principio deve essere applicato a tutti i Paesi nei quali ci sono iscritti fuori dall'Unione europea. Noi pensiamo che, al di là delle tecnicalità, sia una questione di volontà politica: se vogliamo agevolare il diritto di voto di questi cittadini, se vogliamo consentire una partecipazione a coloro che sono sempre italiani, ma si trovano fuori dall'Unione europea, pensiamo che ci siano i tempi necessari per approvare questa modifica di legge. D'altronde, secondo voi sembrava impossibile anche consentire il voto agli studenti residenti all'estero: è una battaglia che come Azione abbiamo portato avanti e vinto. Avremmo voluto dare la stessa facoltà anche ai lavoratori, ma così non è stato. La nostra battaglia pertanto va avanti, noi pensiamo che sia una disparità di trattamento inaccettabile, che i tempi per varare un emendamento che consenta a questi cittadini di votare nei consolati e nelle ambasciate sia qualcosa di estremamente agevole, quindi tocca a voi a voi consentire ciò che ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, ovvero che le prossime elezioni sono una pagina bianca e a scriverla devono essere gli elettori. Ecco, consentiamo anche agli italiani residenti al di fuori di un Paese dell'Unione europea di poter scrivere quella pagina.

Signora Presidente, signor Ministro, il decreto legislativo n. 187 del 2016, all'articolo 6, ha previsto la realizzazione sul territorio nazionale del servizio Numero unico di emergenza europeo 112. Il numero unico per le emergenze funziona secondo il modello della centrale unica di risposta al 112, nel quale vengono convogliate le linee del 112, 113, 115 e 118. il servizio 112 in diversi Paesi europei già rappresenta il modello unico di servizio per le emergenze; l'art. 1, comma 2, della decisione del 1991 recita: "Il numero unico europeo per chiamate di emergenza viene introdotto, ove opportuno,

Ministro, nel nostro Paese è disponibile il sistema di *advanced mobile location*, grazie al quale, laddove non c'è copertura (nemmeno Internet), parte il messaggio SMS, che dà anche la geolocalizzazione; nel momento in cui, invece, si chiama il 112, l'operatore non è sempre in grado di localizzare le persone questo provoca ritardi e, soprattutto nel caso in cui ci sono minori o persone non in grado di dare la loro posizione, si perde tempo. Ora, signor Ministro, quasi 500.000 persone si trovano in questa situazione ed è evidente che conoscere la posizione esatta di chi chiama e la dislocazione sul territorio dei soccorsi limitrofi in quel momento potrebbe aiutare chi aiutare chi opera i soccorsi a reagire rapidamente salvando le vite umane. Eppure, già il Ministro dello sviluppo economico nel 2009 prevedeva il servizio di geolocalizzazione, che risulta ovviamente fondamentale. La geolocalizzazione delle chiamate di emergenza doveva essere introdotta nel nostro Paese già nel 2020, ma ad oggi, in molti casi, le centrali del 112 non sono in grado di utilizzarla. Se a questo aggiungiamo che il numero degli addetti al 112 è calato drasticamente, Ministro, e soprattutto che la qualità degli operatori è scemata, è evidente che andrebbero aggiornati e rivisti completamente i modelli con cui si diventa operatore. Le notizie di cronaca, anche recenti, ricordano impietosamente come la gestione intempestiva delle chiamate d'emergenza e la mancata localizzazione determinano spesso esiti fatali. Non a caso, nella puntata della trasmissione televisiva «Le Iene» dello scorso 31 ottobre 2023 è stato dedicato un servizio a questa problematica con testimonianze e dati allarmanti. Si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente porre porre in essere ai fini del superamento di tutte le criticità descritte, con particolare riguardo all'introduzione della localizzazione immediata ed automatica delle chiamate, all'assunzione di personale specializzato, ai dati del tempo di risposta media nelle varie Regioni e alla riduzione drastica dei tempi di attesa e di invio sul posto dei soccorsi.

- modello, quello italiano, che voglio ricordare è stato riconosciuto nel 2015 come miglior progetto europeo in argomento - è operativo in 15 Regioni con 20 centrali uniche di risposta, servendo circa 43 milioni di abitanti, con una copertura pari a circa il 73 per cento della popolazione nazionale. L'attivazione della centrale unica di risposta avviene sulla base di protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione incaricata dell'attuazione del modello sul proprio territorio, mentre la funzionalità del servizio è regolata da un disciplinare tecnico-operativo che, in linea con le normative comunitaria e nazionale, assicura l'efficacia della gestione delle chiamate di emergenza in un sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale. La centrale effettua la raccolta integrata e coordinata delle chiamate di emergenza a favore delle sale operative degli enti responsabili della gestione e del soccorso e il servizio, nel corso del 2023, ha gestito oltre 21 milioni di telefonate, garantendo altresì la localizzazione del chiamante, il supporto multilingue, la gestione delle chiamate in accesso in accesso equivalente per i cittadini con disabilità, la gestione dell'*eCall* e il monitoraggio delle *performance*. Venendo agli asseriti disservizi, evidenzio che non risultano essere state applicate sanzioni di alcun tipo da parte dell'Unione europea in relazione ad eventuali disfunzioni o mancate introduzioni tecnologiche nei servizi di emergenza. In Italia ogni chiamata di emergenza riceve normalmente una risposta di poco più di sette secondi, con tempi complessivi di gestione della chiamata in linea con il disciplinare che prevede la risposta da parte delle centrali entro dieci secondi. In merito all'inoltro delle chiamate di soccorso da parte della centrale alla sala operativa dell'ente che gestisce l'intervento, da approfondimenti svolti al fine di riscontrare criticità recentemente segnalate anche da articoli di stampa, è emerso che la gestione delle richieste di soccorso avviene in conformità con le modalità operative e le tempistiche previste dallo stesso disciplinare. Relativamente agli operatori delle centrali, tale aspetto compete alle Regioni che si impegnano a reclutarli e a formarli secondo un apposito modulo riguardante compiti e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio, garantendo l'omogeneità dei livelli formativi sul territorio nazionale. Per quanto attiene, infine, al tema della localizzazione del chiamante, il relativo servizio è oggi sviluppato nella maggior parte dei territori in modalità automatica. Al fine di migliorare il sistema di localizzazione, è stata adottata dal Ministero dell'interno anche una soluzione parallela basata sul sistema AML a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non alternativa a quella già in uso, e che in presenza di alcune condizioni è in grado di individuare la posizione puntuale dei dispositivi mobili maggiormente diffusi restringendo la ricerca ad alcune decine di metri. Infine, sempre in un'ottica di ulteriore sviluppo tecnologico, informo che, in attuazione del regolamento n. 444 del 2023 della Commissione europea, è stato avviato un percorso evolutivo finalizzato alla completa digitalizzazione del servizio numero

Le posso assicurare che io stesso ho dovuto usufruire del numero 112: per due rapine in quindici minuti ho impiegato quasi tredici minuti per avere una risposta. Il problema non è ovviamente localizzato in una sola Regione, ma è trasversale in tutta Italia, quindi non sono soddisfatto per quanto da lei detto. Non sono soddisfatto per la mancata implementazione delle tecnologie ancora oggi non esistenti. Non sono convinto e non sono soddisfatto neanche per dover dare molteplici spiegazioni all'operatore prima di poter essere passato al numero necessario, che poi fa perdere ulteriore tempo. Ricordo che nel caso di un codice rosso, i secondi fanno la differenza. Dovrebbe esistere quindi anche il parallelismo con il numero 118, perché potrebbe dare ulteriori aiuti. Ricordo ancora che c'è un numero mancante di persone in servizio nelle Forze dell'ordine che in realtà non vanno a integrare il corpo dei Carabinieri e quello della Polizia. Mancano ancora infatti 20.000 uomini e donne nelle Forze dell'ordine.

Signor Presidente, signor Ministro, si registrano ancora con troppa frequenza, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, episodi di aggressioni a capitreno, controllori e passeggeri da parte di gruppi e individui che vengono fermati perché sprovvisti di titolo di viaggio o perché colti a danneggiare i convogli o le stazioni ferroviarie. In particolare, treni e stazioni sulla tratta Torino-Cuneo-Ventimiglia o Torino-Savona sono spesso utilizzati anche da piccoli spacciatori per i loro traffici. La stazione ferroviaria di Fossano di Fossano (Cuneo) occupa una posizione strategica sulla linea Torino-Savona ed essendo il punto d'origine della linea per Cuneo, necessita di un presidio stabile da parte delle Forze dell'ordine. La stazione di Fossano è il centro nevralgico per i collegamenti ferroviari della Granda, in cui transitano quotidianamente migliaia di passeggeri. È stata pianificata, ormai da diversi anni, la creazione di un posto operativo della Polizia ferroviaria, per garantire la necessaria sicurezza ai cittadini. Negli scorsi mesi si è tenuto presso l'ufficio coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia l'esame congiunto sulla costituzione anticipata del posto di polizia ferroviaria di Fossano, in cui è emersa l'importanza dell'apertura del presidio di polizia nel territorio cuneese, con una pianta organica che consenta un orario di servizio idoneo soprattutto ad assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura. La ristrutturazione dei locali idonei per ospitare il nuovo posto di Polizia ferroviaria è terminata nel mese di marzo 2024 ed anche l'allestimento, allo stato attuale, risulta pronto per ospitare il nuovo presidio. La direzione centrale di sanità ha provveduto in questi ultimi giorni anche a designare il medico competente per le ultime verifiche. Signor Ministro, le chiediamo con la presente interrogazione quale sia la data prevista per l'apertura stabile del presidio di Polizia ferroviaria presso la stazione di Fossano, come sia costituita la pianta organica prevista sin dall'apertura e quale orario di servizio sarà adottato per assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura. PRESIDENTE.

l'onorevole interrogante anche in altre occasioni ha richiamato l'attenzione del Governo, si inserisce nel contesto di un più ampio disegno finalizzato a potenziare la presenza delle Forze dell'ordine nei luoghi pubblici ad elevata concentrazione di persone. Con l'ultima legge di bilancio abbiamo infatti rafforzato la presenza dei militari nelle stazioni ferroviarie, finanziando un'aliquota di personale dedicato di 800 unità. Abbiamo inoltre incrementato il contingente dei militari dell'operazione Strade sicure, portando a 6.000 le unità rispetto alle 5.000 originariamente previste. Contestualmente, la realizzazione sistematica di operazioni interforze cosiddette ad alto impatto, avviate da gennaio 2023, sta producendo risultati positivi in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità, contribuendo ad incrementare la sicurezza e la vivibilità delle nostre città. Dall'inizio dell'anno al 15 maggio scorso, sono stati effettuati nelle città interessate complessivamente ben 501 servizi. Di questi, 178 si sono svolti presso le stazioni ferroviarie e le aree limitrofe, con il controllo di circa 97.000 persone, di cui 151 arrestate e 1.102 denunziate. denunziate. Sempre in questi ambiti, le attività poste in essere hanno portato all'adozione di provvedimenti di espulsione per 116 cittadini stranieri in posizione irregolare, mentre 209 sono state le misure di prevenzione personale complessivamente disposte. Ciò posto, l'ufficio di polizia ferroviaria di Fossano in provincia di Cuneo sarà operativo a partire dal prossimo 3 giugno. Infatti, concluse le attività di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato, e di allestimento degli uffici e degli alloggi collettivi, sono state programmate per i prossimi giorni le verifiche di idoneità dei locali ai sensi della normativa vigente. La dotazione organica del posto di polizia prevede, a regime, ventuno unità complessive, di cui cinque ispettori, sovrintendenti e undici assistenti agenti. Concludo dicendo che, per dare inizio all'operatività del presidio, è prevista una prima assegnazione di undici operatori subito, con orario di servizio articolato sull'arco temporale dell'intera giornata. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Bergesio, *(LSP-PSd'Az)*. Signor Ministro, l'attivazione di questo posto di Polizia ferroviaria rappresenta una risposta concreta non solo alla città e a tutti i fossanesi, ma a tutta la provincia di Cuneo e, me lo lasci dire, agli utenti del trasporto ferroviario piemontese. È una risposta che va a colmare un vuoto che si era creato in passato e soprattutto sul tema della sicurezza la ringraziamo. Siamo sicuri che l'impegno da lei preso in questa autorevole Aula, soprattutto con la sua attività quotidiana, sarà sicuramente mantenuto e rispettato, cosa che per noi è motivo di grande soddisfazione. La gratitudine, signor Ministro, della gente della mia terra va oltre a quello che ci ha confermato oggi. La nostra gratitudine è verso tutte le Forze dell'ordine per il lavoro svolto quotidianamente. Abbiamo visto, proprio in questi giorni, che un pericoloso estremista islamico, autore di violente aggressioni, è stato espulso e rimpatriato in Marocco. di origine marocchina, lo scorso anno si era reso responsabile, in provincia di Cuneo, di una violenta aggressione ai danni di due persone. A ottobre, sempre quest'uomo, dopo aver chiesto un passaggio in auto al vicino di casa, aveva aggredito sia lui sia il figlio disabile. Successivamente, dopo essere sceso dall'auto, aveva colpito anche varie altre automobili di passaggio urlando «Allah akbar». Per bloccarlo erano intervenute, naturalmente, le Forze di polizia. Io da quest'Aula mi permetto di ringraziare, intanto, tutti gli agenti di polizia che svolgono quotidianamente la loro attività, il questore della provincia di Cuneo, il prefetto, il tribunale, la procura e il Ministero da lei diretto, perché siete intervenuti attivando questa espulsione così importante. Il nostro Gruppo da sempre chiede una giusta risposta a questi delinquenti e soprattutto condanne certe per i reati di cui queste persone si rendono colpevoli.

*(FdI)*. Signor Presidente, signor Ministro, i recenti fatti di cronaca a Lambrate e a Milano in particolare evidenziano la sempre più pressante esigenza di interventi decisi e decisivi non non solo per fermare gli sbarchi, ma anche per incrementare i rimpatri dei migranti che non hanno titolo per rimanere in Italia e in particolare di quelli pericolosi per la sicurezza dei cittadini. Il Governo, fin dal suo insediamento, ha messo in campo una serie di misure per aumentare i centri per i rimpatri, per migliorare l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento forzoso, anche incentivando la cooperazione con i Paesi di origine, e per assicurare procedure di ingresso regolare controllato, unico antidoto ai mercanti di morte. Come recentemente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni, l'andamento dei flussi dei migranti irregolari verso l'Italia in significativa diminuzione dimostra che il lavoro in corso sta portando a risultati da valutare con fiducia. Una ulteriore importante linea di azione va dedicata ai rimpatri volontari, assistiti, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni internazionali impegnate in questo ambito. Anche il recente aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale va nella nella stessa direzione e costituisce un altro tassello del cambio di passo delle politiche governative, volte a gestire con pragmatismo ed efficacia il fenomeno migratorio. Tutto ciò premesso, si chiede di sapere quali risultati siano stati conseguiti con le misure già intraprese e quali eventuali ulteriori iniziative siano in via di realizzazione per ridurre la presenza dei migranti irregolari sul territorio nazionale,

Signor Presidente, consentitemi innanzitutto di rivolgere un affettuoso pensiero al vice ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino, a cui intendo manifestare nuovamente la gratitudine mia personale e del Governo per quello che ha fatto e per come lo ha fatto, augurandogli di riprendersi al più presto. Dall'inizio dell'anno sono giunti sulle nostre coste 18.550 migranti, a fronte dei 45.507 dello stesso periodo dello scorso anno, con una diminuzione pari a circa il 60 per cento, come riportato anche dai recenti rapporti di Frontex. Siamo in presenza di un oggettivo segnale positivo, frutto di precise linee di intervento che il Governo ha messo in atto per contrastare il vergognoso traffico di migranti e favorire l'immigrazione legale. Questo si deve, sul versante internazionale, alla collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori, secondo gli indirizzi e le iniziative assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri. Lo scorso 2 maggio ho incontrato i Ministri dell'interno di Algeria, Libia e Tunisia, per consolidare un processo di dialogo regionale nel Nord Africa con l'obiettivo di coordinare gli sforzi per presidiare più efficacemente le frontiere nell'area del Sahel e implementare i rimpatri volontari assistiti. A tal fine ho peraltro istituito al Viminale un'apposita cabina di regia, che si è riunita proprio nella giornata di ieri, anche con la presenza dell'Organizzazione Martedì scorso a Tirana ho partecipato alla Conferenza ministeriale dei Balcani, per rinsaldare la cooperazione in materia di sicurezza e flussi migratori in quel quadrante geografico particolarmente strategico. avvio in Albania delle strutture dedicate alle procedure accelerate di frontiera e al trattenimento dei migranti costituirà un modello innovativo nel contrasto all'immigrazione irregolare, cui guardano con interesse altri Paesi europei. Sul piano dei rimpatri di coloro che non hanno titolo a rimanere in Italia, segnalo che dall'inizio dell'anno al 14 maggio sono stati effettuati 1.779 rimpatri, in aumento rispetto ai 1.681 dello scorso anno, ancorché i rimpatri (CPR) esistenti non siano pienamente funzionali a causa dei continui atti vandalici posti in essere dagli stessi stranieri che vi sono trattenuti. Il 70 per cento dei rimpatriati è transitato dai CPR, sicché ribadisco che è necessario realizzare nuove strutture sul territorio nazionale, comprese quelle dedicate alle procedure accelerate di frontiera, in attuazione del piano straordinario di cui al decreto-legge n. 124 del 2023, in corso di definizione, e contestualmente ripristinare la piena funzionalità di quelli già esistenti. Voglio evidenziare l'importanza di tali strutture ai fini del trattenimento dei soggetti pericolosi, la cui libera circolazione sul territorio nelle more del rimpatrio rappresenta un rischio concreto e attuale per la sicurezza delle nostre comunità. tra le migliaia di persone rimpatriate nel 2023, sono stati eseguiti 77 provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza nazionale, per rischio di radicalizzazione o estremismo, e che dall'inizio dell'anno in corso sono state eseguite 34 espulsioni proprio proprio per gli stessi motivi. Come ricordato dall'onorevole interrogante, è di questi giorni l'inserimento nella lista dei Paesi sicuri di altri sei Stati, tra cui il Bangladesh, il Perù e l'Egitto, che consentirà di fare ricorso alle procedure accelerate di frontiera introdotte dal cosiddetto decreto Cutro anche per i migranti provenienti da tali Paesi e di velocizzare i tempi di accoglimento o di rigetto delle istanze ai fini del successivo rimpatrio. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Balboni,

di un'immigrazione incontrollata e senza alcuna regola non sia un destino obbligato. La sinistra per tanti anni non ha fatto altro che varare norme su norme penso soltanto al cosiddetto decreto Lamorgese, approvato a pochi giorni dalla fine del Governo Conte-*bis* - che praticamente sancivano un principio secondo il quale chi riusciva in qualche modo a mettere piede sul territorio nazionale aveva la ragionevole certezza di poterci rimanere, anche se non aveva rispettato le regole. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in particolare, ha il grande merito di aver convinto l'Europa a considerare i confini dell'Italia come i confini dell'Europa. Chi arriva clandestinamente in Italia arriva in Europa. La strada giusta è quella degli accordi con i Paesi di transito e di provenienza. La strada giusta è quella dei rimpatri veloci. La strada giusta è quella di fare in modo che chi ha dimostrato di essere pericoloso per la sicurezza e per l'ordine pubblico venga trattenuto e rimpatriato. Il dato che lei ha fornito, in base sono stati trattenuti nei CPR sono poi stati effettivamente rimpatriati, è importante, che può e deve essere certamente migliorato, ma che dimostra come chi si oppone alla realizzazione dei CPR non faccia certamente l'interesse dell'incolumità pubblica. Un'ultima notazione, signor Ministro: anche lei ovviamente ne sarà a conoscenza, ma pochi giorni fa la Corte costituzionale ha sancito che il reato di immigrazione clandestina è conforme alla conforme alla nostra Costituzione e alle regole comunitarie. Noi dobbiamo, da un lato, rimpatriare chi arriva senza averne diritto e senza poter invocare la protezione internazionale e, dall'altro, impedire che siano

nonostante le regole e le leggi italiane, perché sappiamo benissimo che queste persone purtroppo, loro malgrado, spesso diventano facile manovalanza per la delinquenza, se non vittime di sfruttamenti che non sono degni

e, ovviamente, a nome di Fratelli d'Italia, mi dichiaro soddisfatto della sua risposta.

delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta di un'interrogazione che riguarda Confindustria Moda, la confederazione di tutte le filiere della moda, una cosa importantissima per l'Italia (parlo di 60.000 imprese,

che era la parte del tessile e abbigliamento, inopinatamente si è ritirata da Confindustria Moda, che era la confederazione di tutti (scarpe, pelletteria, occhiali, accessori e pellicce). Si era riusciti, negli anni intorno al 2016-2017, a mettere tutti insieme, improvvisamente un pezzo, quello principale, si è ritirato. Questo creerà un problema per la nostra filiera della moda, perché ovviamente noi diciamo sempre che non riusciamo a fare sistema, lì si era fatto. Ho quindi chiesto al ministro Urso di farci sapere se fosse al corrente di questa gravissima defezione di Sistema Moda Italia, se sapesse cosa era successo, se avesse delle soluzioni e se fosse intervenuto presso Sistema Moda Italia, Italia, anche con una *moral suasion*. Insomma, è una cosa molto importante. Questo Governo parla tanto di *made in Italy* e poi, quando succede una cosa così grave sul *made in Italy*, non se ne sa niente (poi magari si fa un liceo al quale nessuno si iscrive). Se il ministro Urso avesse la bontà di rispondermi dopo tanti mesi, gliene sarei grato.